ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento. La nuova composizione delle Commissioni, in vigore dalle ore 13 di domani, mercoledì 13 ottobre, è pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna. Come già preannunciato questa mattina alla Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni, nella nuova composizione, sono convocate domani per procedere alla loro costituzione, secondo i seguenti orari, al fine di consentire la partecipazione al voto ai senatori presenti in più Commissioni:

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 21 ottobre. Oggi pomeriggio sarà discussa la relazione della 14a Commissione permanente sui rapporti tra Commissione europea e Parlamenti nazionali. In base ai tempi già ripartiti, il dibattito si concluderà entro questa sera con il voto della risoluzione proposta dalla Commissione o di altro strumento. Domani mattina, alle ore 10, il Ministro della difesa renderà un'informativa sui più recenti sviluppi della situazione in Afghanistan. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi, secondo una ripartizione dei tempi più ampia rispetto a quella per prassi riservata alle informative. Si passerà poi, sempre nella seduta antimeridiana di domani, alla discussione del documento recante la Decisione di finanza pubblica, che proseguirà nel pomeriggio, per concludersi nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 14 ottobre. La seduta antimeridiana di domani avrà termine alle ore 12,45, per consentire la convocazione delle Commissioni permanenti, ai fini del loro rinnovo, come già ricordato. Dopo il voto della risoluzione afferente alla Decisione di finanza pubblica, nella mattina di giovedì prossimo si passerà - ove possibile - al seguito dell'esame del disegno di legge di riforma della professione forense. Le sedute della prossima settimana saranno principalmente dedicate alla discussione di tale provvedimento. Al riguardo, i Capigruppo hanno convenuto sull'esigenza di assicurare al prosieguo dell'esame la dovuta continuità, nell'auspicio di una sua conclusione entro la fine della prossima settimana, anche senza procedere a una formale ripartizione dei tempi. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre l'esame di ratifiche di accordi internazionali. Nella seduta pomeridiana di giovedì 21 ottobre, alle ore 16, il sottosegretario Bertolaso renderà un'informativa sulle conseguenze dell'alluvione che ha colpito il Messinese nell'ottobre 2009, cui seguiranno interventi dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a trattare un argomento di grande rilievo: la Relazione annuale 2009 della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali. E quando dico di grande rilievo, intendo sia sotto il profilo del contenuto sia sotto quello del metodo. Parto dal metodo, paradossalmente, perché non solo la 14a Commissione ha votato una risoluzione all'unanimità, ha anche fatto richiesta della discussione in Aula, con una procedura che non è esattamente consueta, ma con cui si vuole da un lato evidenziare l'importanza di quello che sta capitando - che è un po' sotto gli occhi di tutti noi, però sotto aspetti più tecnici sì, come è giusto, che il Parlamento si riappropri di un ruolo di proposta e di discussione che sembra essere il modo migliore per tagliare qualunque tipo di polemica rispetto all'espropriazione dei poteri del Parlamento stesso. Quindi, quale occasione migliore del confronto in Aula per un processo profondamente innovativo? argomento di grande rilievo sotto il profilo del contenuto, perché questa discussione è un'occasione importante per fare il punto sulla fase ascendente del diritto dell'Unione europea, sui rapporti con i Parlamenti nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea e, soprattutto e specialmente, sul ruolo che ha il Senato della Repubblica. A ciascuno di noi non sfugge che la novità significativa del Trattato di Lisbona è la creazione di un rapporto istituzioni dell'Unione europea-Parlamenti nazionali che non viene più mediato dai rispettivi Governi. Quindi, i Parlamenti nazionali diventano attori del processo legislativo europeo e, grazie a questa novità, acquisiscono un ruolo più significativo e importante. Però, trattandosi della Relazione che riguarda il 2009, è evidente che dobbiamo fare un passo indietro, e questo fa riferimento al periodo intercorso tra la bocciatura del Trattato costituzionale operata da Francia

un dialogo diretto con i Parlamenti nazionali, attraverso quella che viene definita la cosiddetta procedura Barroso, sui cui esiti si concentra proprio la Relazione che oggi andiamo ad esaminare, perché, come dicevo, la relazione è del 2009. Quindi, a differenza di di quanto accade adesso, non si può dare conto della procedura di sussidiarietà che è stata introdotta dal Trattato di Lisbona. D'altra parte, tutti noi sappiamo che tale Trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 e la nuova Commissione si è insediata il 10 febbraio 2010.

perché ci fanno capire quali sono le linee di tendenza rispetto alle quali si è mossa la Commissione e anche come il Senato della Repubblica italiana sia stato in particolare sintonia con questi comportamenti. Nel 2009 i Parlamenti hanno inviato 250 pareri alla Commissione rispetto ai 200 del 2008: quindi, con un aumento significativo del 25 per un dato positivo per tutti i Parlamenti, ma soprattutto per il Senato della Repubblica, perché, permettetemi, il primo elemento che poi ci ha portato con un po' di orgoglio a voler affrontare questi argomenti anche in Aula è che con 17 pareri il nostro ipotetica graduatoria della frequenza dei contributi dati al processo legislativo europeo, si situa al quarto posto sulle 40 Camere dei 27 Paesi. Per capire meglio ciò di cui ci si occupa dobbiamo però guardare da vicino questi numeri. Dei 250 pareri trasmessi, 139 riguardano documenti della Commissione, solo 10 sono stati oggetto di commenti da almeno quattro Assemblee (questa è la soglia minima che viene ritenuta rilevante dalla Commissione europea per approfondire in maniera più specifica i singoli pareri). La cosa che colpisce di questi 10 documenti è che comunque il Senato della Repubblica si è pronunciato sul Programma di Stoccolma, sulla direttiva sull'assistenza sanitaria trasfrontaliera, sulla direttiva sui diritti dei consumatori, sulle decisioni quadro sulla tratta degli esseri umani e sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. Ciò significa che si è mostrata un'ottima capacità di intuire i *dossier* al centro del dibattito politico dell'attività legislativa europea e ciò ha permesso,

si registra una forte concentrazione su temi particolarmente delicati e che nell'ordine sono: lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; la sanità; la protezione dei consumatori; i trasporti e l'energia; l'istruzione e la cultura; l'ambiente e le imprese.

ha rilevato come in meno del 10 per cento dei casi (quindi, in meno di 25 casi) fossero state sollevate questioni di sussidiarietà (ed anche questo, visto in prospettiva rispetto all'evoluzione del Trattato di Lisbona, è un elemento importante) ha ribadito in maniera precisa e puntuale come il meccanismo di controllo della sussidiarietà e il dialogo politico costituiscano due facce della stessa medaglia. E ritengo che il senso del percorso che noi dobbiamo compiere

Ovverosia, in soli sei mesi del 2010 abbiamo espresso un numero di pareri superiore a quello espresso in tutto il 2009.

ma anche grazie alla collaborazione di tutti i commissari che hanno avuto un atteggiamento costruttivo, alla capacità di gestione, alla disponibilità al dialogo da parte della Presidente - che tengo a ringraziare

il rispetto rigido del termine delle otto settimane, non solo perché vogliamo essere europei, ma perché il rispetto del termine di otto settimane (divise fra quattro settimane assegnate alla 14ª Commissione, due alla Commissione di merito ed altre due, eventuali, per una doppia deliberazione) ci dà la

dibattito nell'Aula del Senato. Rispettare il termine di otto settimane significa rendere nota la posizione del Senato prima dell'avvio dei negoziati tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio. Significa essere in grado di garantire con incisività l'azione del Parlamento italiano. È questa la scommessa a cui ci dobbiamo dedicare, soprattutto perché ci troviamo in una fase di transizione, una fase di passaggio fra la procedura Barroso e i nuovi elementi apportati dal Trattato di Lisbona. Dobbiamo creare le condizioni perché tutti quanti insieme si riesca, diventando consci di queste potenzialità, a trasformarle in atti.

ed è la modalità con cui vengono selezionati i progetti legislativi in vista della loro trasmissione ai sensi del Protocollo sulla sussidiarietà. Questo dato emerge, più di tante parole, in maniera estremamente chiara dai numeri.

Di questi 141 progetti, 20 sono stati trasmessi sulla base dei Protocolli di Lisbona: e 20 su 141 è numero assolutamente esiguo.

di secondaria importanza: ad esempio, la proposta di decisione sul servizio europeo per l'azione esterna o la proposta di regolamento sul diritto di iniziativa dei cittadini europei sono passate con la procedura Barroso e vengono analizzate dal nostro Senato grazie a quella

stato infatti introdotto un duplice sistema di esclusione per cui la Commissione, da un lato, sembra decisa a trasmettere solo i progetti legislativi attinenti a settori di competenza concorrente o attività di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri, dall'altro introduce, invece, un elemento di esclusione di tutti quegli atti che costituiscono mero adempimento diretto delle disposizioni previste dal Trattato di Lisbona. Questo significa che non si tengono in considerazione tutto ciò che c'è a valle e le possibilità di interferenza con il processo legislativo di quello che avviene a valle: il rischio è quello di deludere le aspettative di partecipazione che il Trattato di Lisbona ha creato. Per questo motivo la 14a Commissione ha approvato, all'unanimità, una risoluzione che contiene un riferimento critico rispetto ai criteri di selezione degli atti da trasmettere ai sensi dei Protocolli. Per questo motivo ritengo che un dibattito come questo serva a indurre anche un momento di riflessione: uscire da una fase sperimentale per andare verso una soluzione a regime che sia rispettosa, nella lettera e nello spirito, del Trattato di Lisbona. queste osservazioni, perché lo facciamo con la coscienza di chi ha svolto il proprio dovere fino in fondo. Citavo prima i numeri: i 18 pareri espressi nei primi sei mesi ci pongono al primo posto nella classifica dei Parlamenti europei. può significare tutto e può significare niente: sono soltanto elementi di riflessione che servono per rivendicare, con orgoglio, che questi risultati si sono ottenuti con il contributo di tutti. Questa, in conclusione, è la riflessione che lasciamo a questa Aula.

Signora Presidente, signor Ministro, la Relazione della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali costituisce un importante strumento di cognizione sul ruolo che i parlamenti dell'Unione stanno acquisendo nelle dinamiche che alimentano la cornice istituzionale dell'Unione europea. Se sino a non molti anni addietro l'Unione europea si caratterizzava, pur con alcune sue particolarità, quale organizzazione di Stati rappresentati esclusivamente dai Governi, oggi dobbiamo prendere atto che, già con il Trattato di Amsterdam ed ancor di più con il Trattato di Lisbona, l'Unione europea non ha più soltanto un'anima governativa che ne determina le azioni, ma anche un'anima parlamentare che si è andata sempre più incrementando. L'anima parlamentare si è andata affermando con il graduale passaggio delle funzioni svolte dall'Unione europea da organizzazione di mercato ad ente sovranazionale alla quale sono stati conferiti, con i vari trattati, rilevantissimi compiti inerenti la vita concreta dei cittadini. All'accrescersi delle competenze dell'Unione in ambiti che tradizionalmente erano stati riservati alla stretta competenza statale si è andata affermando, quasi a contropartita di tale estensione, l'accrescersi dei poteri della famiglia dei Parlamenti, con in testa naturalmente il Parlamento europeo, che da ultimo con il Trattato di Lisbona si vede riconosciuta una competenza da codecisore nelle delicatissime materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Trattato di Lisbona ha accresciuto anche il ruolo dei Parlamenti nazionali che, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, si sono visti attribuire alcuni limitati poteri, soprattutto in punto di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione. Dal 1° dicembre 2009 i Parlamenti nazionali dell'Unione europea hanno un loro ruolo nell'ambito dell'architettura istituzionale e molti di essi, tra cui senz'altro il Senato della Repubblica, lo stanno svolgendo con grande partecipazione e convinzione.

europeo del 15 e 16 giugno 2006 che, prendendo atto dell'interdipendenza tra il processo legislativo europeo e quelli nazionali, ha invitato la Commissione a prendere in debita considerazione le osservazioni dei Parlamenti nazionali, Dal mese di settembre 2006 ha quindi avuto inizio la trasmissione delle proposte legislative e dei documenti di consultazione ai Parlamenti nazionali direttamente da parte della Commissione europea (la cosiddetta procedura Barroso), con quella effettuata da ciascun Governo nazionale. Sulla base di questa procedura molti Parlamenti hanno cominciato ad esaminare sistematicamente tutti i progetti di atti normativi dell'Unione al fine di far conoscere alla Commissione europea il loro punto di vista

con orgoglio, visto il contributo determinante che il nostro Senato ha fornito sin dall'inizio alla procedura Barroso. Occorre chiedersi le ragioni di questa partecipazione attiva del Senato. Sono essenzialmente due, a cominciare dal fatto che un aspetto importante di questa procedura è stato l'impegno assunto dalla Commissione europea non solo di dare seguito ad eventuali commenti e osservazioni inviati dai Parlamenti sulle singole proposte legislative, ma di replicare per iscritto agli stessi. Ne abbiamo avuto prova anche recentemente perché su risoluzioni inviate dal Senato alla Commissione europea ci sono state risposte da parte della stessa Commissione che indicano questa stretta correlazione. Signora Presidente,

come ha molto ben illustrato il senatore Marino, oggi l'Aula del Senato è chiamata, da un lato, ad una valutazione critica e analitica di un'esperienza, quella del 2009, e, d'altro lato, anche a dare delle indicazioni per il futuro sul punto centrale che è alla nostra riflessione, cioè i rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (per quanto ci riguarda il nostro Parlamento). Insomma, una tappa di quel percorso di cui si è ancora sottolineata da parte del senatore Marino e della collega Germontani la novità politica enorme della partecipazione dei Parlamenti nazionali nella fase cosiddetta ascendente, cioè nell'assunzione della decisione legislativa da parte della Commissione. Il fatto che si tratti del 2009, e quindi di un anno sperimentale (come hanno già spiegato, e non mi soffermo, i colleghi che mi hanno preceduto), ancora fuori dalla procedura del Trattato vero e proprio, ma riferentesi alla cosiddetta procedura Barroso, non deve far sottovalutare l'importanza dell'atto che compiamo nella nostra discussione e nella successiva votazione

queste criticità sono evidenziate, in particolare il metodo di selezione da parte della Commissione delle materie da sottoporre alla procedura

che invece hanno ricadute pesantissime nel vincolare la sovranità nazionale - dall'acquisizione del parere preventivo.

e al rigore con cui le ha seguite che non - mi permetto di dire - a una diffusa e penetrante consapevolezza in tutto il lavoro del Senato e dei senatori. Questo dobbiamo saperlo, nei confronti di alcuno, ma come una consapevolezza politico-istituzionale di quest'Aula. Se la Commissione è riuscita a lavorare in questo modo si deve sicuramente al clima che la Presidente ha saputo instaurare, ma anche alla grande buona volontà dei Gruppi che la compongono e, se mi si permette ancora di più, al senso di responsabilità e all'europeismo conseguente del Partito Democratico e degli altri Gruppi di opposizione. Lo voglio sottolineare, perché sarebbe stato fin troppo facile per noi, cara Presidente, impedire il rispetto dei

dove c'è un problema di costruzione dell'Unione sulla base di alcuni valori. Desidero sottolinearlo, a riconoscimento del valore della Commissione, ma anche dell'opzione politica

Adesso sarebbe stato il momento di portarlo in Aula: non si fa, e temo che per questa legislatura non si farà, e toccherà ancora alla 14ª Commissione svolgere il ruolo di supplenza.

dei bilanci degli Stati. Ebbene, noi andremo a discutere il documento finanziario come fosse un piccolo aggiustamento contabile, senza sapere cosa dirà il ministro Tremonti

sono lieta di intervenire, nella mia veste di Presidente della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, sulla Relazione annuale 2009 della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali.

introdotta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, nel suo Protocollo n. 2, costituisce uno sviluppo non secondario di implementazione della cosiddetta fase ascendente, ovvero della progressiva partecipazione dei Parlamenti nazionali all'elaborazione del diritto comunitario. In altri termini, con il nuovo Trattato viene attribuita ai Parlamenti nazionali, di diritto, la possibilità di inserirsi, in maniera fattiva, nel processo di formazione delle leggi dell'Unione europea. Orbene, il fatto che questa sera discutiamo di tale innovativa funzione dei Parlamenti nazionali costituisce, a mio avviso, un'opportunità da non perdere, in quanto ritengo che l'intero Senato, ossia tutti i 321 senatori dovrebbe essere pienamente consapevole di questa opzione, che ci permette di intervenire, nell'arco delle ormai famose otto settimane, nella definizione *ex ante* di regole che, successivamente, saranno introdotte nell'ordinamento italiano. Proprio a questo proposito, mi preme sottolineare l'importanza precipua della nostra funzione: solo se saremo in grado di fornire il nostro contributo competente nella fase ascendente, avremo poi, in fase di recepimento, la possibilità di trasferire in maniera più efficace e celere, quelle norme dell'Unione europea che ormai disciplinano la vita quotidiana dei nostri cittadini. Se così non facessimo, rischieremmo di vederci "cadere dall'alto", in maniera passiva, tutta una serie di regolamentazioni sulle quali non abbiamo potuto dire alcunché nel momento della loro formazione. Al riguardo, devo rilevare che il Senato della Repubblica, nel suo complesso, ha dimostrato di avere, in termini sia quantitativi che qualitativi, una grande capacità di proposta nei confronti della Commissione europea. Come è ben evidenziato nella Relazione presentata dal senatore Marino, e nella relativa risoluzione approvata dalla 14a Commissione con il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari (che ringrazio fin da ora, ma lo farò ancora nel corso del del mio intervento), occorre riconoscere che in Senato si è instaurato un "circolo virtuoso" che ci vede essere (com'è già stato ricordato) tra le prime Camere dei 27 Paesi membri dell'Unione nell'esercizio del controllo di sussidiarietà e proporzionalità dei progetti comunitari.

Se si va, infatti, a consultare l'elenco delle risoluzioni approvate dal Senato, a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si può desumere che lo scrutinio di sussidiarietà è andato disseminandosi tra tutte le diverse Commissioni permanenti, non rimanendo un'esclusiva prerogativa della Commissione da me presieduta. Per favore, scusate! (Lo dico io e non la Presidente). Si tratta di un fenomeno di non poco rilievo, e da accogliere con assoluto favore, verificatosi anche nella scorsa legislatura, ma che ha registrato una significativa impennata nel corso dell'attuale, come può evincersi come può evincersi dai dati forniti dagli uffici nell'apposito *dossier* in distribuzione. Questo ruolo di «apripista» del Senato mi induce a svolgere un'ulteriore riflessione nella previsione di una futura ed auspicabile revisione della nostra Carta costituzionale in senso federalista e di valorizzazione delle istanze regionali e locali. Il coinvolgimento della nostra Camera nella fase di elaborazione della legislazione comunitaria dovrà essere opportunamente collocato in un sistema che veda lo stesso Senato quale organo costituzionale di raccordo di raccordo tra le realtà regionali e l'istituzione sovranazionale rappresentata dall'Unione europea. In altri termini, a mio parere, il Senato dovrà porsi come snodo essenziale nel canale di collegamento tra le istituzioni di Bruxelles e i nostri territori. Solo in questo modo, infatti, potremo come *decision maker* assolvere al compito irrinunciabile di avvicinare l'Europa ai cittadini, di trasformare, in altre parole, il tecnicismo molto spesso arido, astratto e dettagliato e, quindi, avulso dalla vita reale, tipico della legislazione dell'Unione europea, in un *corpus* di leggi che recepiscano le esigenze vitali di chi vive l'esistenza di tutti i giorni. A tale proposito, vorrei mettere in risalto come, per quanto riguarda la 14a Commissione, sia stato possibile realizzare realizzare determinati risultati anche grazie alla particolare strutturazione interna dei propri lavori. Oltre alla tradizionale Sottocommissione per la fase discendente, presieduta dalla senatrice Licastro Scardino, la Commissione si è articolata anche in una Sottocommissione per la fase ascendente presieduta dal relatore della risoluzione, senatore Mauro Maria Marino. Ritengo che questa si sia rivelata una scelta vincente, in quanto ci ha consentito di esaminare praticamente tutti gli atti comunitari inviatici dalla Commissione

non richiedono una trattazione da parte della Commissione in sede plenaria, con ciò permettendo di vagliare i progetti comunitari che solo apparentemente potrebbero sembrare di minore rilievo. E non posso non ringraziare anche tutta la struttura, i funzionari della Commissione, ma anche tutti i componenti del Servizio degli affari internazionali e dell'Ufficio

di prendere in esame tutte le proposte comunitarie di fase ascendente è stata, secondo noi, assolutamente fondamentale. Abbiamo deciso di esaminare anche quelle che potrebbero sembrare delle minuzie, delle bagatelle, ovvero i progetti che introducono nella normativa comunitaria eminentemente regole tecniche o specialistiche, o che comunque non presentano particolari problemi sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, abbiamo notato che, comunque, la Commissione europea in diverse occasioni ha ripetutamente fatto sapere di apprezzare e raccogliere anche le segnalazioni positive che provengono dai Parlamenti nazionali. In secondo luogo, ci tengo in modo particolare a sottolineare come si sia rivelata proficua l'ulteriore opzione di non limitare lo scrutinio ai soli parametri della sussidiarietà e della proporzionalità, ma di estendere tale giudizio anche ai rilevanti profili di merito di ogni proposta comunitaria. Anche al riguardo ci soccorre, infatti, il punto di vista espresso più volte dalla Commissione europea, che ha dichiarato come i profili di sussidiarietà e proporzionalità siano inscindibilmente connessi al merito delle disposizioni emanate attraverso una data proposta dell'Unione europea. Proprio tale inevitabile inscindibilità ci ha indotto, fin dall'inizio, a svolgere un lavoro che non può essere che onnicomprensivo, ossia che prende in considerazione allo stesso tempo gli aspetti collegati, oltre che naturalmente alla sussidiarietà e alla proporzionalità, anche al merito e, ad esempio, molte volte, anche alla base giuridica di emanazione

Mi riferisco a quel «ruolo sostitutivo» che le viene espressamente conferito dall'articolo 144, quinto comma, del Regolamento e che le consente, qualora la Commissione di merito cui è stato assegnato un atto comunitario in sede primaria non si sia pronunciata o non intenda pronunciarsi, di esprimersi come organo di ultima istanza. Rimarco che la Commissione politiche dell'Unione europea assolve ad un compito cruciale, quasi di chiusura del sistema istituzionale del Senato, che vede garantita in ogni circostanza la facoltà di esprimere la propria voce in Europa. Voglio ricordare che, proprio lo scorso 5 ottobre, il Presidente del Senato ha deciso di incardinare, presso la Giunta per il Regolamento, il documento conclusivo elaborato da un apposito comitato ristretto proprio per aggiornare il Regolamento del Senato al Trattato di Lisbona. Concludo focalizzando quanto detto in premessa. È cruciale per il Senato essere parte attiva e propositiva nella fase ascendente, pena l'irrilevanza in Europa. L'Unione europea è una realtà ultradecennale e consolidata. Non si può mettere la testa sotto il tappeto e far finta che si possa regolare i conti con essa in un secondo momento, quando i giochi nelle varie trattative comunitarie sono stati fatti. Si può aspirare a contare qualcosa in Europa e a dare un contributo sostanziale solo se si è presenti e se si partecipa: altrimenti, è già troppo tardi. Questo, tengo a dirlo, avendo sempre a mente un approccio «di squadra» con il nostro Governo nazionale: nei *dossier* comunitari, il Parlamento e l'Esecutivo devono cercare di agire in via preventiva e di conserva, stringendo anche maggiori rapporti con i nostri rappresentanti del Parlamento europeo, con le Regioni e con il tessuto produttivo e culturale del Paese. Quello che voglio dire è che dobbiamo essere capaci di realizzare un sistema Italia. Sapete la Commissione ha aperto un'indagine conoscitiva per verificare il grado di efficacia, ma anche, purtroppo, le manchevolezze, del sistema Italia in Europa. In conclusione, potrei riassumere il mio punto di vista con una sorta di imperativo categorico: per contare in Europa bisogna esserci! Ed esserci significa, per quanto riguarda noi parlamentari, giocare fino in fondo la carta della fase ascendente ed essere capaci di fare sistema con il Governo, con le altre istituzioni coinvolte e, naturalmente, con i nostri cittadini. Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, dedicare i lavori della nostra Assemblea alla discussione sul tema dei rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali su come i Parlamenti nazionali possano effettivamente e attivamente contribuire al buon funzionamento dell'Unione dovrebbe rappresentare un'occasione e un'opportunità di straordinario valore. Credo infatti che a nessuno possa sfuggire la portata di una condivisione piena e responsabile di tutto il Senato del processo di consolidamento dei rapporti tra Commissione europea e Parlamento nazionale, perché è dalla capacità di muoversi all'altezza di questo ruolo che dipenderà il rafforzamento del Parlamento italiano e il suo essere parte sempre più attiva e consapevole dell'architettura comunitaria. È quindi un segnale di attenzione e di sensibilità importante, da parte della Presidenza del Senato, l'aver voluto cogliere positivamente la richiesta unanime della 14a Commissione di aprire in Aula una discussione in merito alla risoluzione presentata e approvata all'unanimità. A partire dalla presidente Boldi e dal collega Mauro Maria Marino (presidente della Sottocommissione fase ascendente), a tutti i colleghi e al prezioso apporto degli uffici, credo di poter dire che abbiamo ingranato la marcia giusta. Ma una discussione sulle politiche europee, sulle forme e i contenuti con i quali l'Europa rilancia se stessa, non può certo rimanere confinata esclusivamente all'interno della 14a Commissione, pena pena il venir meno di quel valore strategico che vogliamo assegnare alle prerogative attribuite ai Parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo. L'ottima relazione del senatore Marino, che opportunamente ha voluto integrare i dati del 2009 con un quadro storico più articolato e con i dati più recenti riferiti all'anno in corso, ci consegna una situazione complessiva molto confortante ed incoraggiante, che è giusto evidenziare con orgoglio. Non riprendo i dati citati, ma è significativo che l'attività della fase ascendente, con i pareri espressi nell'ambito della procedura Barroso e della procedura di sussidiarietà, ha portato il Parlamento italiano - ed in particolare questo Senato - a collocarsi al primo posto tra i Parlamenti dell'Unione europea per quantità di contributi. Mi preme però sottolineare che non si tratta solo di un dato quantitativamente rilevante da ascrivere nella categoria degli adempimenti formali tecnico-burocratici; si tratta soprattutto, visto l'esame e gli approfondimenti delle singole proposte e visti i pareri inclusivi anche di osservazioni di merito, della qualità del lavoro svolto, che riesce così a coniugare il meccanismo di controllo della sussidiarietà con quello del dialogo politico quale canale essenziale nel rapporto tra Commissione europea e Parlamento nazionale. Da qui la scelta di pronunciarsi su tutte le proposte e non limitarsi esclusivamente a quelle in cui risulterebbe un'eccezione di sussidiarietà. Del resto, su alcuni dei pareri espressi, grazie alla qualità ed incisività dei loro contenuti, la Commissione europea ha posto una particolare attenzione, come si evince dal tenore delle risposte. Oggi però, come è stato detto nella relazione, deve essere anche il momento della riflessione su come uscire dalla fase sperimentale di transizione; su come rendere sempre più incisiva ed efficace l'azione dei Parlamenti nazionali; su come superare definitivamente quel «deficit democratico» di cui soffre il processo di integrazione europea; su come avvicinare l'Europa ai cittadini. Cominciamo però da noi, dall'assunzione di una maggiore e migliore consapevolezza politica - come ha giustamente osservato la senatrice Adamo - dell'impegno cui siamo chiamati con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Credo pertanto sia giusto rimarcare l'esigenza che anche le Commissioni di merito, che già stanno lavorando bene, procedano in modo ancora più sistematico e tempestivo all'esame degli atti e documenti dell'Unione europea,

del perseguimento dell'obiettivo sancito dal Trattato di Lisbona di rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo dei Parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi Governi, debba essere assicurata una presenza più assidua del Governo nelle Camere per riferire sui provvedimenti in discussione in Europa e sulle posizioni assunte nell'ambito delle diverse fasi dell'*iter* legislativo europeo. Di estrema rilevanza è la preoccupata critica avanzata nella risoluzione rispetto ai criteri di selezione degli atti che la Commissione europea trasmette ai Parlamenti nazionali, criteri che sottraggono ai Parlamenti anche atti di grande rilievo, con il rischio perciò di vanificare proprio quel rapporto tra Commissione e Parlamenti e quel potenziamento della partecipazione democratica che stanno alla base del Trattato. Le considerazioni contenute nella risoluzione oggi alla nostra attenzione siano perciò strumento di riflessione comune su cui lavorare nel confronto con gli altri Parlamenti e con la Commissione, per contribuire a superare talune difficoltà ancora presenti dopo la prima fase di rodaggio. Infatti, come ha opportunamente sottolineato il presidente della Repubblica Napolitano, «ci sono forti ragioni di urgenza perché il rodaggio non sia lungo e, soprattutto, appaia presto chiara la direzione in cui ci si intende muovere. La direzione di un più deciso rilancio dello spirito comunitario e della prospettiva dell'integrazione; o la direzione del tradizionale gioco degli equilibri e dei compromessi intergovernativi?». Del resto, le vicende di questi ultimi mesi hanno fatto prepotentemente tornare di attualità il concetto di Europa, la necessità di attuare il processo di integrazione. Quelle vicende ci chiedono di abbandonare definitivamente ogni forma di scetticismo verso il progetto europeo, ogni tentazione di rispondere ai problemi con la chiusura ed il ripiegamento sull'esclusivo egoismo nazionale o locale, ogni diffidenza. Per questo, colleghi, quella di oggi è una discussione importante, ma non riduciamola allo spazio di questi pochi brevi minuti: perché la questione centrale alla quale dobbiamo rispondere va ben al di là dei semplici meccanismi tecnici e delle architetture istituzionali; perché sono occasioni come queste a dover fissare obiettivi più alti e ambiziosi, spetta proprio al Parlamento il compito di indicare tali obiettivi e trovare risposte all'altezza della posta in gioco. Scriviamo insieme una pagina di buona politica. Signor Presidente, cari colleghi, come illustratoci dal relatore, la relazione della 14a Commissione a conclusione dell'esame della Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, mette in luce i risultati eccellenti conseguiti dal Senato e dal nostro Parlamento nel meccanismo di dialogo instaurato fra Parlamenti nazionali e Commissione europea nella fase della produzione normativa comunitaria. Il numero di pareri trasmessi a Bruxelles, ma soprattutto la qualità degli stessi, che si caratterizza non soltanto per valutazioni formali sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, ma anche per l'incisività delle valutazioni di merito nei progetti di legge europea, rende il nostro Paese fra i migliori a livello europeo. E tale dato non può che aumentare, come è stato accennato, con le novità apportate (e già operative da un semestre) da parte del trattato di Lisbona. Infatti il numero dei pareri emessi in questi primi sei mesi di Lisbona supera già quello complessivo realizzato nel 2009. Questo è frutto di un lavoro attento da parte della Commissione 14a, nonché delle altre Commissioni di merito che via via collaborano con noi, dei funzionari di Commissione e della Presidente della stessa, la quale veramente di cuore per tutto quello che sta facendo per rendere alto il lavoro svolto dalla 14a Commissione), la quale ha impostato una direzione efficiente e critica, sapendo valorizzare al meglio le opportunità conferite al nostro Parlamento dal nuovo Trattato. Vorrei quindi ringraziare per il prezioso lavoro di tutti. Non posso poi che concordare con l'osservazione critica che la Relazione in discussione contiene: aver limitato, da parte della Commissione europea, i progetti normativi inviati al nostro vaglio ai soli concernenti settori di competenza concorrente, escludendo quelli di competenza esclusiva europea e quelli che costituiscono adempimento diretto di disposizioni previste dai Trattati, Trattati, ha limitato il numero e la rilevanza delle disposizioni su cui ci siamo potuti esprimere. I dati parlano infatti di soli 20 progetti trasmessi al Parlamento italiano, contro i 141 varati dalle Istituzioni comunitarie. Questo comporta il rischio di perdere una risorsa che la stessa Commissione europea riconosce come preziosa, ossia il supporto dei Parlamenti nazionali, utile come campanello d'allarme per comprendere quali saranno le posizioni degli Stati membri rappresentati in Consiglio dai Governi nazionali, nonché per migliorare,

su cui i Parlamenti degli Stati membri si sono più pronunciati siano stati quelli attinenti materie delicate come lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la crisi finanziaria ed economica e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Questi sono i temi che toccano più da vicino i cittadini e quindi, di conseguenza, i Parlamenti nazionali che li rappresentano. Credo quindi sia utile sottolineare come la Commissione europea non dovrebbe avvalersi di interpretazioni letterali e restrittive del Trattato per limitare il meccanismo di dialogo sulla sussidiarietà, ma dovrebbe all'opposto ampliare tale sfera: difatti, finché non vi sarà una cittadinanza europea consolidata e sentita dai cittadini di Italia, Francia, Germania, Romania finché non vi sarà di conseguenza un Parlamento europeo veramente responsabile politicamente davanti a questi elettori, finché non si creerà un continuo dialogo con una opinione pubblica europea strutturata e capace di far sentire la propria voce, sono proprio i Parlamenti nazionali che devono e possono conferire quella democraticità e sensibilità alle istituzioni europee che manca. Credo che la Commissione dovrebbe allora davvero sfruttare al massimo gli strumenti di dialogo con noi, e non chiuderli. Inoltre non possiamo non sottolineare l'altro aspetto fondamentale che regola il dibattito fra i Parlamenti nazionali e le istituzioni europee: qual'è l'impatto che i nostri pareri e le nostre osservazioni riescono poi a sortire realmente nel processo di formazione del diritto comunitario? È importante riuscire a comprendere, in sostanza, quanto e come può un parere emesso da uno o più Parlamenti nazionali modificare l'assetto iniziale

Valori, una voce al futuro popolo europeo: è infatti l'unica via per un'Europa davvero partecipata e democratica. Auspicando che il suggerimento possa essere trasmesso a livello europeo, esprimo ancora una volta soddisfazione per i risultati conseguiti che la relazione puntualmente fedelmente riporta. Ringrazio per la seconda volta - e non sarà l'ultima nel corso di questa legislatura - la presidente Boldi. *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la risoluzione che siamo chiamati ad esaminare si riferisce, com'è noto, ai contenuti della Relazione annuale per il 2009 della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali.

della Costituzione europea e considerato che i Parlamenti nazionali hanno ora, nel contesto dell'Unione, un ruolo importante. La risoluzione si pone infatti come un'istantanea, una foto dei rapporti realizzati all'interno dell'Unione nel settore legislativo, cogliendone gli aspetti positivi e proponendo le linee di azione per minimizzare quelli meno favorevoli. Ed allora, scorrendo il documento e valutando gli elementi che la risoluzione ci offre, scopriamo una realtà che già percepivamo. Il Parlamento nazionale nel suo complesso e il Senato in particolare si pongono, per numero di atti trasmessi dopo la valutazione di competenza, ai vertici dei risultati che evidenziano l'interazione legislativa con le istituzioni comunitarie nel 2009. Segno, questo, di un continuo coinvolgimento delle strutture parlamentari e di una forte predisposizione dei membri del Senato, senza distinzione di parte, ed in particolare della Commissione preposta alle politiche dell'Unione europea, europea, nei confronti di un'attività considerata di primaria importanza per l'Italia. Scopriamo ancora che la collaborazione del Senato italiano nei confronti delle istituzioni europee si configura non come atto formale, ma come partecipazione attiva e fortemente propositiva. Una partecipazione che mira a rappresentare all'Europa la visione nazionale delle problematiche e a fornire osservazioni e spunti di riflessione, perché quelle istituzioni sovranazionali ne tengano conto (e possibilmente le recepiscano), nel rispetto del ruolo più incisivo che ai Parlamenti nazionali è assegnato. Scopriamo infine che il termine delle otto settimane per l'espressione di un parere definitivo sui provvedimenti che sono sottoposti all'attenzione del nostro Senato è rigidamente rispettato, anche attraverso il frequente ricorso della 14a Commissione alla funzione sostitutiva in caso di assenza di parere da parte delle Commissioni di merito. E questo avviene quale consapevole e ricercato potenziamento del dialogo politico tra l'Italia e le istituzioni europee. Quindi una foto che non può non renderci soddisfatti. Ma, a mio parere, il risultato non poteva essere diverso da quello, molto positivo, che è stato conseguito. Il contributo dell'Italia alle relazioni con le istituzioni europee non poteva non avere un così alto livello, se si considera come l'idea dell'Europa unita sia stata fortemente propugnata nel passato e negli ultimi decenni da tanti personaggi italiani di grande spessore culturale e capaci di lungimiranti visioni politiche; e considerato anche come quell'idea dell'Europa, divenuta concreta attuazione nel secolo trascorso, sia riuscita a coinvolgere fortemente e in larghissima misura la popolazione italiana. Ma la risoluzione della 14a Commissione su cui siamo chiamati ad esprimere un giudizio ha il merito di evidenziare anche aspetti che meno corrispondono alle aspettative italiane di partecipazione attiva alla costruzione europea. Emerge, infatti, un'area - quella dei provvedimenti di legge su materie di esclusiva competenza dell'Unione - che non registra l'auspicata partecipazione dei Parlamenti nazionali. Al riguardo, non è sempre condivisibile, da parte del nostro Paese, il mancato coinvolgimento nel controllo del principio di sussidarietà di progetti legislativi che formalmente incidono in settori di competenza esclusiva dell'Unione, ma che comportano comunque rilevanti conseguenze nei settori di competenza concorrente nazionale. È auspicabile pertanto - e la risoluzione bene lo mette in evidenza - una riflessione congiunta con le istituzioni europee e i Parlamenti degli altri Stati membri per pervenire ad una soluzione che possa meglio salvaguardare gli interessi nazionali in materie che, pur al di fuori dei settori di competenza concorrente, affrontano tematiche comunque d'interesse dei Parlamenti nazionali. Per queste ragioni, per la puntuale sottolineatura del contributo italiano al funzionamento dell'Unione, ma anche delle aspettative che il nostro Paese legittimamente vuole rappresentare all'Europa, la risoluzione al nostro esame merita una convinta approvazione. È un'approvazione che sancirebbe ancora una volta la propensione dell'Italia alla costruzione dell'Unione europea e che concretamente costituirebbe un ulteriore passo verso una dimensione che vedrà il nostro Paese impegnato in futuro nei numerosissimi settori che ci stanno particolarmente a cuore, quali la costruzione di una vera politica estera comune, la realizzazione di Forze armate europee, uno sviluppo sostenibile e sicuro, e tanti altri ugualmente rilevanti.

uno dei problemi più significativi, nell'accidentato cammino dell'Unione europea, è rappresentato dal deficit, percepito come tale dalle pubbliche opinioni continentali, di autentica e dispiegata legittimazione democratica del suo modello istituzionale e dei suoi meccanismi di funzionamento operativo. Ciò è divenuto tanto più cruciale ora, nel mezzo del drammatico guado della "grande crisi", perché l'insufficienza di una risposta opaca o burocratica - o, peggio, di un rattrappimento tecnocraticamente autoreferenziale - dell'Unione avrebbe effetti laceranti sulla credibilità dell'intero processo dell'unificazione. La "grande crisi" ha infatti insieme mostrato la centralità del ruolo propulsivo degli Stati nazionali e l'inadeguatezza di tale ruolo se non sia integrato in coerenti politiche europee (il caso, a maggio di quest'anno, della stabilizzazione della crisi greca mercé lo *special purpose vehicle* è paradigmatico). In coerenza con il recente atteggiamento italiano, va dunque rafforzato, nella medesima direzione di valore e secondo lo stesso "orizzonte di senso" della *soundness* democratica, il progressivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. L'Italia sta robustamente facendo la sua parte con la piena adesione alle procedure di dialogo tra Parlamento nazionale e istituzioni europee e in particolare con la procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. Il formidabile *score* del nostro Senato (primo assoluto nel 2010), ricordato dall'amico relatore Marino, è molto chiaro. Il meccanismo di controllo dei Parlamenti nazionali sul rispetto del principio di sussidiarietà è stato da subito interpretato dal Senato nel senso più ampio, come ha voluto appropriatamente ricordare la nostra presidente Boldi. La nostra interpretazione poggia su una duplice convinzione: da un lato, sull'utilità di esprimersi su tutte le proposte legislative sottoposte alla procedura, anche quando non si rilevino profili critici; dall'altro, sull'impossibilità, nel valutare la sussidiarietà, di prescindere dalla proporzionalità, dalla base giuridica e dal contenuto di merito della proposta. Questa interpretazione, che non si discosta dall'impostazione della medesima Commissione europea,

Io credo sia importante sottolineare come l'impegno del Senato nel rapporto con le istituzioni europee sia improntato anche al pieno coinvolgimento del Governo. A proposito, ministro Ronchi, sulla distorta vicenda del trilinguismo brevettuale tenga duro, siamo assolutamente con lei. Il nostro dialogo diretto con la Commissione europea non intende collocarsi in una condizione di estraneità o addirittura di ostile intrusività rispetto all'azione del Governo, ma anzi, si propone come un propellente o almeno come un supporto alle posizioni negoziali italiane, per rafforzare la loro efficacia nei confronti di Bruxelles. Parlamento e Governo devono farsi da sponda in questo per cercare di creare finalmente un vero «sistema Italia» che sia in grado di far valere e di offrire il suo grande patrimonio nazionale all'Europa. In questo senso, ad esempio, è da intendersi il noto «emendamento Boldi-Santini» (entrato in vigore come articolo 4-*quater* alla legge n. 11 del 2005) sulla «partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà», che non a caso ribadisce con nitidezza il vettore dell'«interesse nazionale» nella sinergia Camere-Governo. Ma anche le altre modifiche apportate alla citata legge n. 11, con l'attivo concorso della maggioranza e dell'opposizione, seguono le stesse tracce. L'auspicio è che sia questa impostazione, di cooperazione attiva e di integrazione propulsiva tra ruolo del Parlamento e ruolo del Governo, a ispirare la preannunciata riforma complessiva della legge n. 11 del 2005, che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Lungo la medesima traiettoria si muove l'indagine conoscitiva della 14a Commissione del Senato, che è stata avviata proprio sul «sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'Unione europea con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria». L'intenzione è quella di individuare gli elementi su cui occorre lavorare per riuscire a diventare punto di riferimento in Europa, aumentando l'influenza della nostra Nazione in un'Europa che deve prendere atto del ritrovato ruolo di protagonista dell'Italia e della sua rinnovata vocazione a guidare il processo, da un lato, di "ribaricentramento" dei tradizionali poteri continentali, dall'altro, del loro collocarsi esplicitamente in una nuova chiave paneuropea e mediterranea.

in modo molto sintetico soltanto per dire che ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito. Emerge chiaramente che questo è stato un dibattito proiettato verso il futuro; così si deve leggere il senso delle proposte venute circa la questione che riguarda il Regolamento (la cui discussione, come evidenziava bene la Presidente, per fortuna è già stata incardinata il 5 ottobre); così è da leggere il circolo virtuoso che si è venuto a creare e che fa sì che in questo momento non ci siano arretrati. Questo è un grande merito degli Uffici e del gioco di squadra che è stato fatto. Soprattutto mi è piaciuto il passaggio in cui si evidenziava che il lavoro che si sta facendo non ha valenza quantitativa ma qualitativa, e questo lo si vede dalla qualità dei pareri e dal dibattito che c'è sia nella Commissione plenaria che nella Sottocommissione nella fase ascendente. Proprio per questo, e concludo,

collaborare per un unico obiettivo. In questo senso, lavoriamo per il futuro.

la Camera dei deputati) di essere sempre più pienamente partecipe di questo grande processo che è il processo decisionale europeo.

e la piena, grande consapevolezza del Parlamento che il proprio contributo ed un coinvolgimento sempre più presente e attivo può dare la possibilità al Paese di incidere con una maggiore efficacia sulla definizione delle politiche cosiddette comuni e sulla elaborazione della legislazione europea.

Quanto più intensa e attenta è la partecipazione alla fase ascendente, tanto più forte, incisiva e reale può essere la posizione del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione. A questo riguardo riporto un esempio. Proprio

la piccola e media impresa italiana, la stessa radice culturale della nostra Italia e, soprattutto, le nostre posizioni all'interno dell'Unione europea. La linea del Governo, dunque, è volta ad elaborare un nuovo approccio dell'Italia all'Europa basato sulle seguenti priorità: rafforzare il coordinamento ed elaborare una visione strategica di difesa dei nostri interessi, degli interessi del sistema Italia; realizzare un vero sistema che possa mobilitare tutte le potenzialità, gli attori e capace di influire nel processo di decisione dell'Europa; migliorare la nostra capacità di attuare la normativa europea e quindi - importante - rispettarne le regole. In questo In questo approccio il Parlamento deve essere - ed il dibattito di oggi lo ha dimostrato in modo inequivocabile - il grande protagonista.

prevedendo che il Governo debba fornire al Parlamento una precisa ed adeguata informazione sui contenuti e sull'impatto di ogni proposta di atto legislativo dell'Unione al fine della valutazione e del rispetto del principio della sussidiarietà.

ho cercato di rafforzare ulteriormente l'interazione tra il Governo e le Camere disciplinando tutti i meccanismi che il Trattato di Lisbona mette a disposizione a disposizione dei Parlamenti nazionali per un loro incisivo, proficuo, costante coinvolgimento nei diversi livelli del processo decisionale della nostra Europa. Tra questi, è certamente significativo il controllo sul rispetto del principio della sussidiarietà. Attraverso pareri motivati, ciascun ramo del Parlamento può trasmettere al riguardo alle istituzioni dell'Unione europea le proprie valutazioni, e può intervenire direttamente nel processo decisionale, vigilando insieme agli altri Parlamenti nazionali sul corretto esercizio, da parte dell'Unione, delle proprie competenze concorrenti. Ritengo, però, altresì importante, e soprattutto particolarmente preziosa per il Governo, la possibilità che avete, come Parlamento, di pronunciarvi sul merito delle proposte di atti presentati dalla Commissione, attraverso atti di indirizzo rivolti al Governo. Mentre, infatti, il controllo di sussidiarietà è destinato ad esplicare i suoi effetti a livello di Unione europea, questa seconda opportunità che il Trattato di Lisbona fornisce esplicitamente ai Parlamenti consente di rafforzare la posizione dell'Esecutivo in uno spirito di squadra, di *team*, destinato a fare finalmente emergere ciò che per troppi anni è mancato, cioè il sistema Italia. Tutto ciò richiede un grande, forte e deciso impegno da parte del Governo, di tutta l'amministrazione e, permettetemi, anche un grande cambio di mentalità.

Signora Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia sulla risoluzione della 14a Commissione,

il dialogo dovrà consentire di avere uno scambio di vedute che non si limiti alle proposte legislative e che vada ben oltre la questione della sussidiarietà. Sono quindi fermamente convinta che l'aver tenuto insieme le varie procedure che si intersecano in riferimento all'esame in fase ascendente possa costituire una pratica parlamentare da continuare in futuro. In tal senso, auspico che la Giunta per il Regolamento, che si è recentemente convocata, segua l'impostazione data dal Comitato coordinato dalla presidente Boldi, relativa all'attuazione in Senato del Trattato di Lisbona. Alla logica della procedura Barroso corrisponde una progressiva esigenza di armonizzare a livello parlamentare le diverse culture giuridiche costituzionali che ancora sussistono nei singoli Paesi membri dell'Unione europea. Ciò vuol dire che la Commissione europea svolge attualmente un significativo lavoro di raccordo istituzionale, fornendo le linee guida di una riforma dei singoli ordinamenti, in modo da superare divisioni e superiorità nazionalistiche. In ultimo, voglio sottolineare che il ruolo dato dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali costituisce una delle nuove frontiere del costituzionalismo contemporaneo. Se si supera il blocco concettuale di chi ritiene che il potere estero degli Stati sia ancora da riservare ai singoli Governi, si potranno apprezzare le molteplici opportunità di azione per i Parlamenti offerte dal loro inserimento nell'architettura istituzionale europea. Non posso poi non fare un richiamo a quanto recentemente affermato da alcuni commentatori circa le innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona. Mi riferisco al fatto che il Trattato Trattato ha, per la prima volta, attribuito ai Parlamenti nazionali una serie di compiti nel procedimento di formazione della legislazione dell'Unione europea. Alcuni di questi compiti sono attribuiti specificatamente, non già ai Parlamenti nazionali ma, trattandosi di Parlamenti bicamerali, a ciascuna Camera di essi. È evidente che i poteri delle Assemblee rappresentative sovrane, ovvero le due Camere, sono disciplinati da una fonte esterna al esterna al circuito costituzionale interno. Per la prima volta i Trattati europei dettano poteri, regole e procedure che valgono anche nei confronti delle istituzioni parlamentari nazionali. Con il Trattato di Lisbona le competenze di Senato e Camera vengono disciplinate da una fonte di un ordinamento giuridico diverso da quello italiano, e le stesse Camere, per quanto riguarda i poteri individuati dal Trattato di Lisbona, sembrano aver perduto la possibilità di decidere sulla loro competenza disciplinata dalla fonte europea. Credo che questa prospettiva dovrà essere tenuta in grande considerazione quando parleremo di riforme istituzionali nel nostro Paese e in particolare del Senato federale. Forse per ora la prima vera riforma costituzionale l'ha fatta proprio il Trattato di Lisbona. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia.

in quanto rappresenta una delle rare occasioni in cui il lavoro, annuale e di grande respiro, di una delle Commissioni del nostro Parlamento entra direttamente nel dibattito dell'Aula plenaria. Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi della 14a Commissione, e soprattutto la presidente Boldi, perché il nostro lavoro, preciso e costante, ha permesso al Senato, al Parlamento italiano, e quindi all'Italia tutta, di detenere il primato per numero e qualità dei contributi inviati alla Commissione europea sulla produzione normativa di Bruxelles. Visto che purtroppo l'Italia si posiziona in cima alle classifiche europee solitamente per ragioni non meritorie, essere per una volta alla vetta della classifica per i risultati positivi conseguiti nel dialogo Commissione-Parlamenti nazionali è davvero una bella soddisfazione. Vorrei dire grazie ancora una volta, quindi, al lavoro di tutti i colleghi di tutti i colleghi della 14a Commissione e alla direzione dei lavori tenuta dalla presidente Boldi, precisa, attenta, puntuale, la quale ha permesso non soltanto di rispettare il termine delle otto settimane per pronunciarsi sulla sussidiarietà degli atti comunitari, ma ha tramite l'impulso conferito con il meccanismo della doppia deliberazione, sollecitato le Commissioni di merito ad adempiere agli obblighi europei nei termini prestabiliti. Credo proprio, su questo punto, che sia importante sfruttare ancora di più il fatto che i componenti della 14a Commissione fanno anche parte di altre Commissioni permanenti proprio per dare una ancora maggiore sinergia al compito di cui siamo stati investiti con il Trattato di Lisbona. Quello che mi preme sottolineare, e che la stessa Commissione ha riconosciuto nella sua relazione, è infatti la circostanza che, nel meccanismo di dialogo con il legislatore europeo, i Parlamenti nazionali, ed il nostro Senato in particolare, non si sono confrontati soltanto sugli aspetti tecnici, ossia la valutazione del rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà sulle proposte di legge europee che ci vengono sottoposte, ma hanno analizzato, apprezzato e talvolta sollevato ad obiezioni critiche la sostanza politica, normativa e sostanziale del progetto normativo. Questo significa che i Parlamenti nazionali non si sentono dei burocrati di Bruxelles, utilizzati solo per salvaguardare disposizioni formali, ma vivono il rapporto con l'Europa in paritaria cooperazione, insistendo proprio su aspetti di merito e non solo di forma. Come ricorda la Commissione, questo significa una precisa volontà: non lasciare che la conduzione del ruolo italiano nelle istituzioni comunitarie si affidi soltanto al Governo, con la rappresentanza e la voce assicurata ad ogni Esecutivo dal Consiglio dei ministri e dal Consiglio europeo, ma sia un indicatore della voglia, per il Parlamento, di contribuire come attore principale nel processo normativo comunitario. Ebbene, credo che anche questo sia un fattore assolutamente fondamentale, da non tralasciare, colleghi: dato che abbiamo assistito in questa legislatura ad un Senato e ad una Camera dei deputati che facevano il ruolo delle comparse nel grande film della produzione normativa, ritrovarle, per una volta, e grazie alla sponda di Bruxelles, attori protagonisti è sintomo che ancora esiste un'area di autonomia e una voglia di fattiva influenza negli affari pubblici da parte del Parlamento; un Parlamento che se non trova un Esecutivo, ed un capo dell'Esecutivo, che gli impone *diktat* normativi a suon di decreti-legge, ha la capacità di esprimersi in maniera consistente e con brillanti risultati. Pertanto, cari colleghi, vi chiedo di non fermarvi qua e di contribuire anche a livello interno per riprenderci la dignità che la Costituzione ci affida: il Parlamento è, come tutti voi sapete, e come purtroppo molti di voi dimenticano sovente, depositario della potestà legislativa che può soltanto delegare eccezionalmente e sotto precisi principi vincolanti, al Governo. Cerchiamo di non dare più deleghe in bianco al Governo, né a livello europeo né a livello nazionale. Partendo dalla riflessione di questo pomeriggio, non possiamo non concludere con una riflessione sugli scenari per il futuro dell'Europa e per il ruolo che gli Stati membri avranno, Governi ed Esecutivo, nelle relazioni intracomunitarie. La Commissione europea e la 14a Commissione hanno richiamato la necessità di far proseguire la Procedura Barroso, ossia il dialogo politico fra Commissione e Parlamenti nazionali, nonché di potenziare quegli strumenti di interfaccia

dunque che il ruolo che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali devono assumersi è fondamentale: solo una spinta all'integrazione, delle norme e delle politiche, che nasca dai Parlamenti democraticamente eletti può portare ad un'Europa rappresentativa e coesa. Pertanto, esprimendo il voto positivo e la soddisfazione dell'Italia dei Valori per i risultati che emergono dalla relazione che dibattiamo oggi, chiudo questo intervento assicurando che l'Italia dei Valori svolgerà il proprio ruolo, che mi impegno a sostenere per un'Italia sempre più europea e per un'Europa sempre più democratica. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel Trattato di Lisbona il ruolo dei Parlamenti nazionali é disciplinato essenzialmente in un articolo specifico e nei due Protocolli allegati al Trattato. Ulteriori disposizioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui principi di sussidiarietà e proporzionalità sono contenute in altri articoli del Trattato. In particolare, il Trattato di Lisbona introduce nel Trattato sull'Unione europea un nuovo articolo 8C, che illustra il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo. La norma prevede che i Parlamenti nazionali contribuiscano attivamente al buon funzionamento dell'Unione. In particolare, i Parlamenti nazionali: sono informati e ricevono i progetti di atti legislativi europei dall'Unione europea; hanno il compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà;

sono informati delle domande di adesione all'Unione europea; partecipano alla cooperazione interparlamentare in ambito europeo. Prima di entrare nel merito del documento in esame, vorrei soffermarmi brevemente su alcuni dati. L'attività del Senato in ambito europeo ha conosciuto negli ultimi anni un forte e costante sviluppo. Mi riferisco all'esame di progetti normativi comunitari e allo svolgimento dell'attività conoscitiva e delle relazioni interparlamentari. Tutto ciò ha reso possibile una maggiore consapevolezza sugli effetti e sulle opportunità dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. L'attività del Senato nell'esame degli atti legislativi e non legislativi dell'Unione europea aveva registrato, nel corso della scorsa legislatura, un un primo forte incremento, che ha portato a concludere l'esame di 26 atti comunitari. Tale dato è stato raggiunto in due anni di mandato e, già dall'esordio della XVI legislatura, l'attività registrò un ulteriore incremento. Questi risultati positivi sono dovuti

Il Senato partecipa - inoltre - a numerosi incontri interparlamentari che si svolgono sia presso il Parlamento europeo sia nel Paese che che detiene la Presidenza dell'Unione europea. Si tratta di una prassi che ha permesso un dialogo strutturato tra parlamentari europei e parlamentari nazionali su temi specifici di attualità. Anche in questo settore si registra un significativo incremento dell'attività del Senato. Ciò premesso, entro nel merito del documento che stiamo esaminando. Esso costituisce, senza dubbio, un adempimento importante, che ci permette di capire quale sia il rapporto che i Parlamenti hanno con l'Unione europea, e soprattutto i rapporti del nostro Senato con le istituzioni dell'Unione europea. La nota nuova da evidenziare riguarda la nascita di un rapporto tra istituzioni dell'Unione e Parlamenti nazionali, non più mediato dai rispettivi Governi. In definitiva, si tratta di un rapporto attraverso il quale i Parlamenti nazionali sono i protagonisti del processo legislativo europeo. I dati forniti dalla Commissione europea, sia per quanto riguarda il quadro generale dei rapporti con i Parlamenti nazionali, sia per quanto attiene al ruolo del Senato, sono molto positivi. Non mi soffermo molto su tali dati in quanto sono stati esposti in maniera esauriente nella relazione della 14a Commissione permanente, redatta dal collega Marino, che precede la risoluzione. Tali numeri dimostrano, che il Senato ha in primo luogo mostrato una grande capacità di cogliere i dossier al centro del dibattito e dell'attività legislativa europea. In secondo luogo, il Senato si è pronunciato su di essi in modo tempestivo e adeguato, esprimendo soprattutto pareri ricchi I documenti selezionati per l'esame dei Parlamenti nazionali riguardano principalmente argomenti quali la sicurezza, la giustizia, l'energia, l'ambiente, i trasporti, le imprese, la cultura. Su tali argomenti il Senato si è trovato perfettamente in linea con le scelte dalla maggioranza dei Parlamenti. In ogni caso - e mi avvio a concludere, signora Presidente la cosa importante da sottolineare è che, con 23 atti esaminati, il Senato si colloca al terzo posto in assoluto per numero di contributi, preceduto solamente dal Senato ceco e dal Bundesrat tedesco. Il Parlamento italiano nel suo insieme, con un totale di 40 contributi, risulta invece essere il primo Parlamento dell'Unione. Per quanto riguarda, infine, gli atti trasmessi dalla Commissione europea nell'anno in corso il Senato è nettamente al primo posto in Europa, avendo dato il suo contributo su 18 di essi. Pertanto, così come è evidenziato nella risoluzione, il mio l'auspicio è che si esca dalla fase sperimentale per arrivare ad una soluzione a regime volta ad intensificare e a rendere sempre più efficace il lavoro dei Parlamenti nazionali. Per tali ragioni, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

alle relazioni tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, approvata lo scorso 21 luglio dalla 14a Commissione, abbiamo avuto un'impagabile occasione per meglio delineare quale effettivo impatto abbia arrecato, nel nostro ordinamento, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Mi preme precisare che, in seno alla Commissione politiche dell'Unione europea, si registra una forte condivisione per quanto riguarda l'impostazione

Paese assumeva delle posizioni esclusivamente filo-comunitarie, soprattutto attraverso declamazioni retoriche o ideologiche, in favore di un'Europa sovranazionale, autoescludendosi così dall'interpretare a pieno le proprie posizioni nell'interesse nazionale. Fra l'altro, nonostante le declamazioni retoriche ed ideologiche e la mancata interpretazione dell'interesse nazionale, il nostro Paese si poneva molto spesso tra tra i primi posti nella *black list* dei Paesi dell'Unione, collezionando un gran numero di infrazioni relative all'attuazione della normativa europea nel diritto nazionale.

ripensare il modo di concepire il collegamento tra i Parlamenti nazionali ed il complesso meccanismo legislativo dell'Unione europea, utilizzando a piene mani le nuove opportunità che ci vengono offerte dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore lo scorso dicembre. A tal riguardo, il nuovo ruolo che ci viene attribuito, cioè il controllo della della sussidiarietà delle proposte comunitarie, deve essere considerato non più, come si pensava un tempo o come ancora oggi ritengono alcuni che vorrebbero perpetuare le modalità del passato, come un appesantimento o addirittura un intralcio all'*iter* di formazione della legislazione europea. Al contrario, la possibilità di esprimere il proprio parere in fase ascendente da parte dei Parlamenti nazionali diventa un fattore di stimolo e di arricchimento nel processo di formazione delle leggi comunitarie. Diventa una prerogativa ed un'occasione fondamentale per il nostro Paese per dare voce alle esigenze ed ai bisogni della nostra gente. Il Parlamento, infatti, oggi vede riconosciuta ed amplificata la possibilità di meglio rappresentare le istanze dei nostri territori, delle nostre popolazioni e, quindi, può meglio assolvere il compito di canalizzare questi interessi presso le istituzioni comunitarie. L'attiva partecipazione del Parlamento può, quindi, contribuire a colmare quel drammatico *gap* che che ancora esiste tra l'Europa e i nostri cittadini: quel deficit democratico che impedisce ai singoli soggetti - consumatori, imprenditori - di comprendere pienamente la ragione delle decisioni che vengono prese a Bruxelles, cioè da un'entità spesso percepita come lontana dai problemi di tutti i giorni. È giunto il momento che i consumatori, gli imprenditori, i soggetti della società civile prendano consapevolezza che l'Europa ha loro dato più voce. A questo proposito, vorrei mettere l'accento sul fatto che, quando la 14a Commissione esprime un suo parere o osservazioni, o pone condizioni su un provvedimento in fase ascendente, si registra sempre di più un fenomeno di assoluto rilievo: la stessa Commissione europea replica con risposte argomentate ai rilievi posti dalla 14a Commissione. La Commissione europea ci risponde anche quando le nostre osservazioni sono meramente non ostative, evidentemente ravvisando la necessità di realizzare comunque un *feedback* con il singolo Parlamento nazionale. Lasciatemi infine esprimere alcune ultime, ma non per questo meno importanti, considerazioni che riguardano la Sottocommissione pareri per la fase ascendente della quale sono componente. Tra i componenti della Sottocommissione si è instaurato un ritmo di lavoro davvero ammirevole, grazie anche al suo presidente senatore Mauro Maria Marino, che voglio qui ringraziare. Voglio anche ringraziare tutto lo *staff* legislativo che ruota intorno alla 14a Commissione

non può essere redatto alcun Resoconto sommario che ne fornisca la dovuta visibilità. Ritengo che sia giunto il momento di accordare, anche alla Sottocommissione pareri, la possibilità di pubblicare un breve Resoconto. La Lega Nord ritiene giunto il momento che il Senato conferisca la facoltà di resocontazione

che hanno il diritto di conoscere, di valutare e di esprimersi in merito. Concludo esprimendo il convinto voto a favore del Gruppo della Lega Nord Padania sulla risoluzione approvata dalla 14a Commissione in merito al documento della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella discussione generale è già stato ampiamente esaminato il merito della risoluzione in discussione; non intendo quindi ripetere quanto già espresso dai colleghi. Userò questo tempo per sviluppare qualche ulteriore breve riflessione. Premetto che, quando si parla di Europa, mi considero un estremista e sono quindi tra quanti hanno ritenuto il Trattato di Lisbona un'occasione per molti aspetti mancata per dare maggiore forza e prospettiva al progetto europeo. Premetto anche - per essere stato testimone diretto delle lunghe ed estenuanti trattative che hanno portato alla sua definizione che sono perfettamente consapevole che i tre passi indietro compiuti da molti Paesi, tra cui l'Italia, in quella occasione hanno almeno consentito a tutta l'Europa di fare un passo in avanti, coinvolgendo nelle decisioni comuni anche le Nazioni e i Governi più recalcitranti. Quando si parla del Trattato di Lisbona bisogna quindi osservarlo con la lente della *realpolitik* ed obbligarsi a vedere il bicchiere mezzo pieno, apprezzando quanto di positivo esso ci propone. Il documento oggi in discussione sottolinea uno degli aspetti più positivi e più significativi che il Trattato di Lisbona ci ha regalato: la definizione di un ruolo da forte protagonista per i Parlamenti nazionali. L'articolo 12 ha rappresentato certamente una delle più interessanti novità inserite dalla Conferenza intergovernativa. Esso persegue e consegue - come ho detto - l'obiettivo ambizioso di rendere i Parlamenti nazionali interlocutori diretti dell'Unione, acquisendo un ruolo formalmente indipendente dal Governo dello Stato membro cui appartengono. Verrebbe da dire, in un periodo in cui la funzione e addirittura l'utilità dei Parlamenti è spesso messa in discussione dagli Esecutivi di alcuni Stati europei (e quello italiano non sembra fare certamente eccezione), che a Lisbona si è scelto di andare contro tendenza, riconoscendo alle Camere di ciascuno Stato membro lo *status* di interlocutore forte, credibile e decisivo. Del resto - come ha ricordato il senatore Mauro Maria Marino - seppure informalmente la Commissione europea dal 2006 aveva già nei fatti adottato procedure e metodologie di lavoro che prevedevano un forte coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, mostrando di nutrire una fiducia nel dialogo politico che merita di essere ricordata, menzionata e, perché no, lodata, soprattutto perché tale metodologia non è stata immune da critiche. Si è parlato da più parti di potenzialità destabilizzanti del cosiddetto meccanismo di *early warning*, così come numerosi commentatori hanno voluto intravedere nel coinvolgimento dei Parlamenti nazionali un elemento di ulteriore complicazione del già complesso processo decisionale europeo. Quanto illustrato oggi in quest'Aula, in particolare dalla relazione del senatore Mauro Maria Marino, dimostra a nostro avviso che invece si può e si deve guardare con ottimismo e con spirito di positiva collaborazione all'attuazione del Trattato di Lisbona e di quanto disposto dall'articolo 12. Certamente la nuova condizione in cui il Trattato pone i Parlamenti impone loro di guardare avanti e di crescere in autonomia ed autorevolezza, accettando ed affrontando sfide più alte ed ambiziose, non ultima quella di contribuire - non lasciando questo compito ai soli Governi - alla scrittura del diritto europeo, non accontentandosi più di intervenire soltanto nella fase del recepimento o della risposta da dare a qualche procedura di infrazione. di infrazione. Fondamentale è comunque il contributo che i Parlamenti hanno già dato e saranno chiamati a dare in misura sempre più significativa nell'esercizio del controllo della conformità dei progetti normativi comunitari al principio di sussidiarietà. Senza addentrarci nei dettagli dei meccanismi introdotti dal Trattato, quello che dobbiamo guardare con attenzione è la sfida di forte significato politico che esso lancia implicitamente ai Parlamenti, ma anche ai singoli parlamentari. In poche parole, le nuove procedure, se da un lato spingono, o addirittura obbligano, le istituzioni europee e i Governi a dialogare con i Parlamenti nazionali, dall'altro incitano i Parlamenti, ma soprattutto i singoli parlamentari, ad interessarsi più assiduamente a quanto accade nelle istituzioni europee e a darsi conseguenti criteri organizzativi, personali e non personali. Secondo alcuni, con l'andare del tempo e il crescere del numero delle iniziative della Commissione poste al vaglio dei Parlamenti, sorgeranno problemi di coordinamento delle Assemblee nazionali. Da questo punto di vista, riteniamo che vada supportata ed aiutata a crescere la funzione di raccordo svolta dalla COSAC, la Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei e comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea. La COSAC può rappresentare in questo frangente il luogo più appropriato per il confronto politico e lo scambio di informazioni sulla sussidiarietà. Per questo, riterremmo utile che, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, si alimentasse una discussione e si avanzassero proposte su come rendere sempre più efficiente tale organismo, e sempre più efficace la partecipazione italiana ad esso. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ministro Ronchi, il Gruppo del Partito Democratico valuta positivamente il contenuto della risoluzione in esame ed esprimerà pertanto il suo voto a favore. *(Applausi dai

signor Ministro, onorevoli senatori, le riflessioni sull'Europa che stiamo svolgendo oggi in quest'Aula, e in particolare sul rapporto tra i Parlamenti nazionali e le istituzioni europee, che è l'oggetto del documento che abbiamo all'esame, danno testimonianza dell'avvio di una fase positiva e costruttiva per l'Unione europea, successivamente al periodo di stallo istituzionale, politico e ideale di qualche anno fa. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore lo scorso dicembre, non ha solo migliorato l'assetto istituzionale dell'Unione, adeguandola alle sue nuove dimensioni demografiche e geografiche, ma ha anche dato nuova linfa e nuovo ottimismo all'idea stessa del nostro stare insieme in Europa. Da questo punto di vista, il maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nei lavori che si svolgono nella capitale dell'Unione, Bruxelles, costituisce forse il cardine di un processo di recupero di credibilità e di consenso nei confronti dell'ideale europeo. Coinvolgere i Parlamenti nazionali significa aprire una finestra di dialogo con le popolazioni dell'Europa; significa non sottrarsi al vaglio critico dei cittadini e dei loro rappresentanti, nella convinzione che ciò non porta ad un indebolimento, bensì a un rafforzamento della coesione politica europea e a un miglioramento della qualità della legislazione che riguarda tutti i cittadini dell'Unione. Questo, signora Presidente, è lo spirito con cui si sta svolgendo questo primo esercizio post-Lisbona del controllo di sussidiarietà da parte del Senato italiano, che ha adottato da subito un atteggiamento di piena adesione alle nuove procedure e al nuovo ruolo che il Trattato ha conferito ai Parlamenti nazionali. Il Senato, e la 14ª Commissione in particolare, si è fatto promotore di un approccio che si è rivelato essere quello più proficuo: un'interpretazione per così dire estensiva delle nuove opportunità procedurali connesse con la fase ascendente della legislazione europea, europea, verso la quale ora anche altre Camere parlamentari in Europa sembrano voler convergere. Un'interpretazione che considera essenziale, anzitutto, esercitare il vaglio parlamentare su tutte le proposte legislative europee che rientrano nella procedura di verifica della sussidiarietà, proprio per sfruttare appieno le potenzialità che questo strumento offre; e che considera, inoltre, che per un compiuto esercizio del controllo di sussidiarietà non sia possibile prescindere dai connessi aspetti concernenti il principio di proporzionalità, la base giuridica della proposta e la disciplina materiale che sostanzia la proposta stessa. In questo senso, la stessa Commissione europea ha affermato che il meccanismo di controllo della sussidiarietà e quello del cosiddetto dialogo politico costituiscono due facce della stessa medaglia e che il principio di sussidiarietà è parte di una relazione politica più estesa tra la Commissione e i Parlamenti nazionali. Ne consegue che limitare l'espressione del parere ai soli aspetti della sussidiarietà in senso stretto, o addirittura ai soli casi in cui dall'esame risulti un rilievo critico sul rispetto del principio di sussidiarietà, significherebbe svilire e svuotare ampia parte di questa relazione politica tra la Commissione e i Parlamenti nazionali. I dati quantitativi che vedono l'Italia, e il Senato in particolare, in vetta alle graduatorie dei pareri espressi ai sensi del Protocollo n. 2 sul controllo di sussidiarietà non richiedono ulteriori commenti. Per questo risultato non si può non dare atto del ruolo svolto in particolare dalla 14a Commissione, strutturata al suo interno con un'apposita Sottocommissione per la fase ascendente (presieduta dal senatore Mauro Marino), ma anche di tutte le Commissioni del Senato, in cui il processo legislativo europeo sta progressivamente assumendo la rilevanza che merita. Tuttavia, a questi dati quantitativi si aggiungono gli innegabili riscontri qualitativi relativi ai pareri espressi nell'ambito di queste procedure, ampiamente testimoniati - come ha ricordato anche il relatore - dal tenore delle risposte della Commissione europea, anch'esse spesso puntuali e molto interessanti, a dimostrazione del fatto che questo dialogo tra il legislatore europeo e il legislatore nazionale non è solo un esercizio formale, ma include aspetti sostanziali di notevole rilievo. In questo senso anche la perplessità, espressa nella risoluzione al nostro esame, relativa alla scelta della Commissione europea di non trasmettere ai sensi dei Protocolli molte proposte che, pur attenendo alla competenza esclusiva dell'Unione, presentano ampie ricadute su settori di competenza concorrente con gli Stati membri, costituisce un valido contributo che il Senato ha l'opportunità di offrire per il rafforzamento dei meccanismi del dialogo tra i Parlamenti nazionali e le istituzioni dell'Unione europea. Dichiaro quindi il convinto voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà

dell'annosa vertenza tra una ditta della provincia di Treviso e l'Agenzia delle entrate.

il presidente della Repubblica Napolitano, dopo aver reso omaggio alla memoria dei caduti sul lavoro e dopo avere espresso la sua solidarietà a quanti hanno sacrificato la propria salute e la propria integrità fisica, deplorando il continuo aumento degli incidenti e delle morti bianche, ha esortato ad un maggior impegno per la prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro, ispirata - cito testualmente - «ad una cultura della legalità e sicurezza e basata su una costante e forte vigilanza sul rispetto delle norme e delle condizioni di lavoro». Condividendo in pieno queste parole, voglio rilanciare la nostra proposta di ripristinare le norme approvate dal Governo Prodi in tema di sicurezza. Oggi purtroppo la tutela della sicurezza e il rispetto dei diritti sul lavoro vengono spesso sacrificati in nome del profitto e dell'arricchimento, ma il lavoro che dà dignità ed assistenza e sussistenza non può diventare svilimento della condizione umana. Il Governo e questa maggioranza prestino ascolto alle parole del Presidente e si cambi rotta, visto che fino ad oggi non hanno fatto altro che smantellare il Testo unico sulla sicurezza con i relativi tagli, e adesso si accingono, con il cosiddetto disegno di legge sulla semplificazione, a dare un'altra spallata alle norme sulla salute dei lavoratori. In più, in questi giorni, signora Presidente, il Ministro del lavoro - è questo il nocciolo del mio intervento - ha prodotto un vergognoso *spot* sulla sicurezza che, invece di esortare le aziende al rispetto della legge, colpevolizza sottilmente i lavoratori con la scusa di responsabilizzarli. Lo *spot* infatti recita: la sicurezza devono pretenderla se si vogliono bene. *Ergo*, come è stato scritto recentemente su un quotidiano, chi cade da una impalcatura, chi muore asfissiato nella cisterna o schiacciato da un trattore ha un problema di autostima? La verità che non viene detta è che l'attuale condizione di lavoro e la diffusione della precarietà non permettono al lavoratore di pretendere nulla, nemmeno il rispetto dei diritti minimi, conquistati dopo anni di lotte sindacali. Per questo, Presidente, ho aderito convintamente ad un appello lanciato da un gruppo di medici del lavoro e di rappresentanti sindacali che chiedono il ritiro di questa pubblicità, e invito l'Assemblea e i colleghi a fare altrettanto.